*relatore*. Signora Presidente, nella relazione introduttiva ho cercato di esporre i punti salienti che sono stati introdotti nel corso dell'esame parlamentare nel disegno di legge presentato dal Governo e mi sono soffermato sulla rilevanza degli stessi. In sede di replica vorrei fare solo alcune considerazioni generali sia di natura metodologica, che sui contenuti.

del Parlamento. I contenuti del dibattito sono stati profondi, l'intento da parte di tutti i senatori costruttivo: la volontà di migliorare il testo della legge, l'autonomia del giudizio, il leale confronto e la leale collaborazione tra maggioranza e opposizione e tra Governo, maggioranza ed opposizione, tutto ciò insomma non può che rendere il relatore e, credo, tutto Parlamento veramente molto soddisfatti. È una prova vera di efficacia ed efficienza del Parlamento,

Credo che anche l'illustrazione ed il voto degli emendamenti continuerà in questo solco, cosicché si giungerà ad una legge sul federalismo che, a prescindere dall'espressione del voto finale, dovrà visto una maggioranza e un'opposizione in grado di entrare nel merito dei contenuti, di confrontarsi e di produrre un buon testo normativo. Ovviamente, le posizioni rimarranno quelle che saranno espresse nel voto sugli emendamenti e in sede di voto finale, ma non vi è dubbio che il testo risente della buona prova e del buon clima che si è instaurato. Sul piano dei contenuti il testo il testo sul federalismo a questo punto si presenta più equilibrato, più definito, più rispettoso più rispettoso del rapporto tra Stato e livelli di governo decentrati, più rispettoso del rapporto tra le Regioni, gli enti locali e lo Stato. delle norme introdotte mi porta a dire che il testo ha superato un vaglio abbastanza severo da parte dei senatori, e lo ha superato positivamente. provvedimento si presenta più equilibrato sotto il profilo del rapporto tra territori; penso all'introduzione del patto di convergenza, alla definizione precisa del carattere verticale della perequazione, all'introduzione delle funzioni fondamentali dei Comuni, alla migliore definizione dei livelli essenziali, dei servizi ai cittadini. Insomma, non c'è dubbio che non si presenta come frutto della volontà di una parte, ma come il testo dell'intero Parlamento e, all'interno di esso, di una maggioranza e di un Governo nel loro complesso.

i territori possono trarre da questa legge lo slancio e lo stimolo a fare meglio e tutti insieme a puntare verso l'alto, in una prospettiva di nuovo sviluppo che parte dai principi fondamentali del federalismo, quali quelli della sussidiarietà e della responsabilità. In questo testo tali principi ci paiono meglio definiti, più precisi e meglio individuati.

adeguatamente introdotta all'interno di questo provvedimento, una perequazione che naturalmente punta a ridurre le grandi divergenze in materia infrastrutturale che ancora esistono nel Paese. Ci sembra insomma di aver posto ulteriori elementi per disegnare una nuova distribuzione di poteri all'interno della Repubblica italiana,

nell'ambito legislativo e che esalta le funzioni amministrative di Province e Comuni. Questo mi pare un altro elemento di grande e significativa rilevanza del testo che questo Senato si appresta ad approvare. Certo, alcune questioni possono essere ancora migliorate. Non c'è dubbio che i dati daranno luogo, nel corso della legislazione delegata - me lo auguro - ad ulteriori miglioramenti e il clima e le strutture che sono state individuate da questo Parlamento certamente favoriranno questo aspetto. Direi che i decreti delegati, avvalendosi dei dati, porteranno a nuove e migliori puntualizzazioni delle grandi caratteristiche che prima mi sono sforzato di delineare.

delle modifiche; se il clima e gli strumenti che abbiamo adottato funzioneranno, così come prevediamo, anche quelle situazioni potranno essere risolte in maniera positiva, ridando slancio - ripeto - all'intera Repubblica italiana.

nuovamente le singole questioni che sono state introdotte se non per ritornare solo ad una di esse, quella riguardante la programmazione pluriennale delle risorse dei fondi di coesione sociale.

più utile per lo scopo a cui quei fondi sono destinati, più utile per le Regioni e per la porzione di territorio italiano a cui sono assegnati. Insomma, non vi è dubbio che possiamo dirci abbastanza soddisfatti e che la maggioranza ha dato prova insieme di grande coesione e di grande apertura, così come l'opposizione ha dato prova di grande capacità di elaborazione e di costruzione insieme all'intero Parlamento. Tutto questo, naturalmente, sotto un coordinamento del Governo che - anche se sono parco in queste manifestazioni - mi consentirete di ringraziare perché ha mostrato particolare sensibilità e spirito di collaborazione con il Parlamento intero. Due ultime osservazioni prima di terminare. Mi piace ricordare che in alcuni punti di principio è stata riprodotta la necessità di un grande semplificazione degli adempimenti, in particolare di quelli tributari. Oggi uno dei problemi dell'Italia è l'espansione della burocrazia; la semplificazione - e non è un caso che il Ministro che si è occupato di questo provvedimento è quello della semplificazione - è una delle ricadute che auspichiamo, altrimenti il federalismo non avrà avuto gli effetti che riteniamo opportuni. I cittadini devono sentire da queste riforme un

fondamentali. Ciò che auspichiamo dal federalismo è anche una riduzione nel tempo della pressione fiscale. Il cittadino questo comprenderà se grazie a tale norme

possano derivare da quei principi di sussidiarietà e responsabilità che abbiamo prima delineato. Queste sono le grandi questioni

Il controllo del Parlamento che sarà particolarmente penetrante - così come previsto dal testo elaborato dalla Commissione - certamente aiuterà

il relatore di maggioranza, senatore Azzollini - che quello di ieri è stato davvero un dibattito inusuale in quest'Aula e di questi tempi. credo che avesse ragione il senatore Mercatali quando ieri ha detto che dovrebbe essere la norma di un Parlamento della Repubblica italiana affrontare grandi problemi come questi con capacità di ascolto reciproco e con la serietà degli argomenti che sono stati portati. Così, però, non è. Pertanto, credo sia giusto segnalare l'inusualità di questa discussione ed il fatto che il metodo seguito rappresenta una rara eccezione nell'avvio di questa legislatura repubblicana. rappresentanti del Governo, che al dialogo e al confronto reale sui temi del federalismo (sul quale rimangono grandi ed importanti punti aperti, su cui poi mi soffermerò) corrisponde l'umiliazione pressoché quotidiana che il Parlamento riceve da parte del Governo, con il reiterato ricorso ai decreti-legge e con un Presidente del Consiglio che non perde occasione per negare qualunqueruolo all'opposizione.

che noi abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare in questa discussione potranno essere compresi dalla grande opinione pubblica italiana. In altri termini, non dobbiamo farci condizionare dalle nostre reciproche posizioni di maggioranza e di opposizione nella ricerca

Il ministro Tremonti, tuttavia, mi può aiutare nel sostenere quelli che per il Partito Democratico e per l'opposizione rappresentano ancora i grandi interrogativi aperti di questa discussione. A potermi aiutare, però, non è il ministro Tremonti del 2009, ma il professor Tremonti del 1994.

Leggo a pagina 65 per arrivare all'imposta che la finanzia (*posterius*), prima si deve definire chi fa che cosa, poi si possono definire gli strumenti fiscali».

Carta delle autonomie locali e federalismo fiscale non possono andare separate, perché non vogliamo dare nuovo carburante ad una macchina vecchia, qual è lo Stato italiano così com'è organizzato oggi. Vogliamo riorganizzare e decentrare

di trovare nel libro di Tremonti del 1994 un riferimento al tema degli scenari e delle proiezioni necessarie per dare una base che il professore di allora ci avrebbe dato ragione. Vediamo se oggi il Ministro ci dà ragione su un altro punto per noi fondamentale, e voglio spiegare bene di cosa sto parlando. Il Governo ha proposto un provvedimento

politicamente al Governo una relazione tecnica che ci indichi, sulla base dei meccanismi attuali della legge, quali sono gli effetti sulla distribuzione territoriale delle risorse.

effettuati anche oltre le regole stringenti del Patto di stabilità. L'ordine del giorno del Senato per quanto riguarda la doverosa restituzione dell'ICI.

serve ad impedire che si fotografi l'attuale offerta di servizi enormemente squilibrata tra le diverse parti del Paese

il traguardo di una buona legge sul federalismo fiscale possa essere raggiunto con il massimo di consenso possibile. Ministro Calderoli, le abbiamo dato più volte atto della sua disponibilità. Ministro Tremonti, la ringraziamo ancora per la sua presenza: non vi nascondiamo che molte delle possibilità di arrivare a questo risultato positivo sono adesso nelle vostre mani.

Signora Presidente, signori senatori, la domanda che mi è stata posta è una domanda sull'impatto economico del testo in discussione. Le variabili che devono essere conteggiate per formulare il calcolo sono un numero elevatissimo e cercherò di rappresentarle. Non sono stilizzabili in formule meccaniche come nei sistemi semplici; mi sono informato per dare una risposta scientifica - un sistema olistico come il corpo umano, interagiscono tra di loro essendo interdipendenti e coniugate. C'è un modo razionale, tuttavia, per rispondere alla vostra domanda, che penso sia una domanda più politica che tecnica, più sintetica che specifica e analitica,

dobbiamo condividere tutti insieme - maggioranza, opposizione e soggetti di governo coinvolti ai vari livelli - la direzione verso cui andare, la direzione di massima e di sistema. Conosciamo i passi che dobbiamo fare lungo quella direzione e ad ogni passo abbiamo chiaro che è fondamentale calcolare prima e calcolare dopo. A questa altezza di tempo possiamo dare (e cercherò di dare) una risposta razionale e procedurale. Credo che sia davvero difficile, ma non per limiti del

L'esercizio che dovremmo fare vede in gioco variabili interdipendenti e coniugate, che si configurano in questi termini: abbiamo dodici tipi principali di tributo in gioco; abbiamo cinque soggetti politici titolari dei cespiti tributari; nel testo che stiamo discutendo e che è stato discusso qui in Senato undici tra criteri e principi istitutivi; tutto è sotto il rispetto di due fondi di sussidiarietà e solidarietà iscritti nella Costituzione della Repubblica; vi sono otto tipi di procedure attuative e un numero non ancora specificato di decreti attuativi. Più analiticamente, i tributi che sono oggetto della delega federale sono IVA, ICI, imposte di registro ipotecarie e catastali, addizionali varie, IPT, RC auto e accise, tributi propri di scopo eventualmente istituiti. I soggetti tra cui deve essere operato l'arbitraggio di potere fiscale e federale sono lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni e gli organi orizzontali di

le politiche di bilancio da costruire con regole coerenti con il Patto di stabilità, l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il superamento del criterio della spesa storica (addizionale e fabbisogno standard), la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, la premialità, la territorialità articolata anche infunzione della conformazione geografica, orografica o della insularità, le forme di fiscalità e di sviluppo compatibili con il sistema comunitario e così via. I fondi di cui ho parlato sono i due grandi fondi istituiti con una logica di unità e di solidarietà nell'articolo 119 della Costituzione. Le procedure e l'*iter* attuativo si articolano in otto forme: i decreti legislativi da adottare dal Governo, la Commissione parlamentare, il parere della Commissione bilancio, il comitato esterno dei rappresentanti delle autonomie territoriali, la commissione tecnica paritetica, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la Commissione di vigilanza sull'anagrafe, eccetera.

caso saranno interattivi e avranno tra di loro effetti compensativi. È difficile quindi simulare l'impatto di un tributo. Ammesso che si arrivi, a valle di tutte quelle complessità, ad immaginare un decreto,

Questo per dire della elevatissima complessità tecnica, che è tipica e propria di un simile congegno. Comparativamente, in tutti gli ordinamenti costituzionali dell'Europa e del mondo i congegni di federalismo fiscale sono ad alta complessità istituzionale

discutendo di altri testi - formulare, a questa altezza di tempo, un esercizio di impatto politico. C'è anche, se volete, una prova del nove di carattere non per sottrarmi ad una domanda assolutamente giusta, ma per prendere l'impegno a rispondere a quella domanda fra un po' di

proprio dell'ordinamento della Repubblica italiana, che le leggi delega devono essere fatte oggetto di analisi economica e, semplificando, di copertura solo se esse stesse producono direttamente effetti economici. Diversamente, se la delega rinvia per l'effetto economico agli effetti propri dei decreti attuativi, che sono l'effetto della delega, il calcolo della copertura e l'analisi di impatto vengono svolti solo sui decreti, non sulla delega.

secondo luogo, ciò non è necessario, essendo la ragione di cautela costituzionale e di controllo politico soddisfatta nell'analisi dei singoli decreti. Cercherò di fare due esempi fortemente indicativi. La legge delega n. 59 del 1997, la legge Bassanini, è stata costruita in questi termini: non c'è stata un'analisi d'impatto economico della legge delega, mentre c'è stata un'analisi d'impatto economico dei decreti attuativi. Ma soprattutto è indicativa la storia costituzionale della legge n. 281 del 16 maggio 1970, la grande legge che istituisce il sistema delle Regioni.

su impugnazione della legge istitutiva delle Regioni fatta da Lombardia e Veneto. In sintesi, la Corte costituzionale, su ricorso attivato contro la legge istitutiva delle Regioni da Lombardia e Veneto, dice che la Costituzione non pone la condizione della verifica dell'impatto finanziario, rimandandola ai criteri legislativi. quindi un meccanismo coerente con quello che ho cercato di dire prima. L'analisi deve essere fatta, è un obbligo costituzionale e in questa sede è anche un obbligo politico che il Governo assume, ma non può essere fatta in base alle sentenze della Corte, correttamente: rappresentando quelle sentenze un principio logico, non può essere fatta *ex ante* sulle grandi deleghe. Lo stesso tipo di considerazioni sul ricorso la Corte costituzionale ha fatto a proposito della legge Bassanini, pure oggetto di ricorso. Per inciso (ma è un inciso costruttivo), faccio notare che il decreto legislativo che attualmente disciplina la finanza regionale non ha un impatto marginale, perché poi quell'unico articolo applicativo, immerso in un decreto *omnibus*, ha modificato tutto il sistema, ha sostituito il vecchio fondo sanitario con una dinamica compartecipazione all'IVA, ha rimodulato l'impianto della perequazione, ha introdotto le addizionali IRPEF.

quelle a cui il Governo è chiamato qui a rispondere (e deve rispondere), seppure in una forma che non può essere attuale ma procedurale.

producono un effetto di rigidità e di non arbitrarietà e quindi, a valle, di ragionevole prevedibilità in linea di massima.

risorse finanziarie di cui stiamo discutendo è previsto nella delega da operare in base al criterio dei costi standard, che dovrebbero finanziare sanità, assistenza, scuola, trasporto trasporto pubblico locale. Se la scelta è quella del costo standard, è evidente che prima bisogna avere il costo standard e poi calcolare il meccanismo finanziario di finanziamento. È difficile ragionare in termini di meccanismo finanziario di finanziamento se non è stato prima definito il costo standard, che è la base da cui partire. - ripeto - il testo di cui stiamo discutendo rispetta totalmente la Costituzione della Repubblica nel suo impianto politico fondamentale di unità, di solidarietà

Un altro punto non marginale dà l'idea di una clausola generale, di un equilibrio di fondo che comunque rappresenta un principio. Nell'articolo 21 del testo d'iniziativa

possibile, ma non corretta, un'interpretazione minimalista di questa regola. L'articolo 21 codifica dentro questo testo un principio costituzionale. Il Patto di stabilità e crescita non è un pezzo a un pezzo a sé di trattato internazionale, è un pezzo della Costituzione vigente della Repubblica. È quella che si può chiamare la Costituzione esterna, ma è pur sempre un criterio costituzionale ed è la dominante sotto la quale è scritto questo testo. Il Patto di stabilità e crescita naturalmente può essere discusso nel suo razionale economico: noi non lo discutiamo e in più lo attuiamo. Formule o ipotesi legislative devianti rispetto a questo schema sono incostituzionali e per noi inaccettabili. Ma questo è un fattore di forte garanzia per dare dare un'idea dell'effetto finale dell'impatto economico del provvedimento. Comunque sia, sta sotto la Costituzione per i criteri di unità e di solidarietà e sta dentro la Costituzione, assumendo che consideriamo costituzionale anche il Patto europeo di stabilità e crescita. Ci sono altri elementi che hanno una rilevanza politica fondamentale per formulare una risposta politica alla domanda sull'impatto. Tutto il testo è articolato e sviluppato nella logica di procedure condivise tra il Governo, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, di procedure condivise tra questi soggetti e anche nelle sedi di fatto costituzionali in essere dentro il nostro ordinamento, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni. prodotto del testo che stiamo discutendo, che ne è la prova: lo spirito politico della discussione che stiamo svolgendo, che è lo spirito di una costruzione condivisa.

in essere da troppo tempo, come è stato rilevato dal Presidente della Repubblica. Anche se non formalmente, sostanzialmente è una legge costituzionale. Sappiamo bene che il fondamento della democrazia è «*no taxation without representation*».

una sede nella quale abbiamo iniziato ad elaborare dati tecnici, avendo assunto l'impegno che deriva dalla profonda convinzione che per realizzare i decreti attuativi servono dati omogenei,

Avere dati non omogenei e non condivisi è come non averli. Stiamo costruendo una base di dati convinti del fatto che sia una ragionevole base di partenza. Abbiamo coinvolto in questo processo le istituzioni tecniche di Governo, dalla Ragioneria abbiamo coinvolto l'ISTAT, l'ISAE, la Banca d'Italia. Siamo aperti ad ogni tipo di contributo in questo campo. Appena avremo i primi flussi li presenteremo. Pensiamo che la discussione possa avvenire solo una volta acquisiti quei dati. Comunque, l'impegno politico è di iniziare a lavorare insieme sui dati per calcolare l'impatto dei decreti attuativi prima di emanarli e di realizzare quel calcolo insieme a tutte le forze politiche o tecniche interessate a tale esercizio.

incontrati sul percorso da chi aveva cercato di intraprendere il federalismo fiscale partendo o dalla spesa storica o dal gettito dei tributi), il cosiddetto uovo di Colombo, è legato alle funzioni - fondamentali e non,

non solo in senso astratto ma con un riferimento preciso ad un costo standard e quindi ad un parametro predeterminato che garantisca efficienza, efficacia e qualità del prodotto,

aumentato. L'aver attribuito un costo standard che necessariamente non può superare il più alto costo rispetto alla spesa storica ci fa desumere che comunque non potrà che esserci un calo

Quindi non c'è possibilità di anarchia dell'aumento della pressione fiscale. Anzi, dovrà esserci un contenimento rispetto a una quantificazione e a una limitazione di quel costo.

la materia concorrente sia per quello che riguarda le funzioni degli enti locali, arriva addirittura a dare quattro definizioni diverse senza una ulteriore specificazione. Di qui la necessità in questo momento di far partire il federalismo fiscale superando il principio del «è nato prima l'uovo o la gallina», cercando di farli partorire insieme,

il primo passo avanti rispetto alla definizione di funzioni, fondamentali e non, da parte dei tre soggetti di governo (Comuni, Province e Regioni) che per la prima volta hanno espresso un consenso unanime su questa proposta. Il Governo si impegna per la settimana prossima a portare in Consiglio dei ministri la Carta delle autonomie locali per poter dare un seguito a quel periodo di transitorietà; in un incontro avuto con il sottosegretario Davico ed il ministro Maroni

ma è altrettanto vero che difficilmente un federalismo fiscale si può realizzare compiutamente in assenza di una ridefinizione di quella materia che è stata già oggetto del lavoro della Commissione affari costituzionali della Camera, quale aveva raggiunto una serie di intese rispetto ad alcuni punti che devono essere modificati e su cui tutti convergono. Mi riferisco alla ridefinizione della forma del Parlamento: una Camera che si occupi degli affari dello Stato, un Senato delle Regioni, la fine del bicameralismo perfetto. Sono tutti interventi su cui il Governo promuoverà un dibattito probabilmente porterà anche una propria proposta di riforma costituzionale che faccia propria l'esperienza della passata legislatura e da lì faccia discendere il resto. Visto che è il Senato quello che viene più modificato rispetto al passato, l'intenzione del Governo è che l'avvio di tale discussione avvenga proprio in questo ramo del Parlamento e non alla Camera, come stava invece accadendo nella passata legislatura.

L'aliquota riservata deve avere una propria flessibilità, così come garantita per le addizionali; deve essere garantita quella progressività che è richiamata all'articolo 53 della Costituzione, che è stato previsto proprio con riferimento a tale aspetto È chiaro che i limiti entro cui occorre muoversi non vengono fissati dalle Regioni: è lo Stato che fissa la manovrabilità di tale aliquota.

- di un federalismo solidale, in cui cioè i diritti civili e sociali definiti dalla Costituzione siano garantiti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo però anche richiesto

l'amministratore dell'ente locale o della Regione trarrà un vantaggio dall'emersione, di conseguenza ne trarrà vantaggio anche lo Stato. Credo molto in questo.

so benissimo riveste un ruolo molto importante, abbiamo accolto la proposta di creare una Commissione *ad hoc* oltre alla Commissione bilancio per gli aspetti finanziari.

compartecipazioni, tributi propri e fondo perequativo devono garantire la copertura integrale delle funzioni pubbliche pubbliche comuni. Questo cosa vuol dire rispetto a dire di no ad alcuni emendamenti che ancora residuano? Non è un no di contrarietà:

ma credo che quando andremo a rivedere anche quelle funzioni dei Comuni dovremo avere molto chiaro che esistono le funzioni fondamentali, le funzioni obbligatorie e un numero indefinito di funzioni

abbiamo seguito la strada, inizialmente proposta dalle Regioni e accogliendo le loro indicazioni da noi modificata, di dare solo sulla parte strutturale, quindi legata al conto capitale, una copertura integrale con riferimento ai costi standard, lasciando la parte della spesa corrente con la perequazione della capacità fiscale.

così come le funzioni transitoriamente utilizzate per definire i costi standard; stiamo ancora in questo momento cercando di giungere ad un testo che possa avere una condivisione dei tre livelli di governo. Mi auguro che

di ogni maggioranza che cambia le regole, ogni volta quella successiva le abrogherà per farne diverse, con buona pace del cittadino cornuto e mazziato. Dimostriamo di essere cresciuti.

finanziario della riforma del federalismo fiscale che non ci appare convincente, pur essendo stata resa con un tono e un approccio che apprezziamo, perché sottolinea la complessità e l'imprevedibilità allo stato delle conseguenze finanziarie della riforma. Il Servizio del bilancio del Senato, come sempre puntuale ed illuminante, ha trattato i profili di coerenza della legge delega di cui stiamo discutendo con l'articolo 81 della Costituzione: sono problemi che rimangono aperti, essendo noto l'orientamento costituzionale in base al quale è il legislatore delegante - e non quello delegato - che deve disporre in ordine alla copertura *ex* articolo 81 della Costituzione. Lei, signor Ministro, ha citato diverse pronunce, tranne quella più significativa e rilevante sul tema: la sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976 che dispone

una serie di osservazioni e dubbi sui rischi di squilibrio finanziario soprattutto nel periodo transitorio, allorquando si potrà verificare l'emanazione di provvedimenti di entrata e di spesa di segno opposto, suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Un tema ancor più rilevante questo alla luce della sintesi che lei, signor Ministro, ha fatto e che vede nel testo 12 tipi di tributi, 5 soggetti pubblici e 11 tra criteri e principi. Il Servizio del bilancio segnala anche la necessità di assicurare la compatibilità delle norme e dei principi di delega con il quadro delle grandezze finanziarie pubbliche ed è questo, a nostro modo di vedere, il tema principale. L'ISAE, l'ISTAT e la Corte dei conti hanno avuto modo, con varie argomentazioni, di evidenziare l'opportunità e la necessità di valutare *ex ante* l'impatto finanziario di una riforma di tale portata. Dalla prima all'ultima seduta delle Commissioni riunite abbiamo sollevato questo problema. È un problema politico che prescinde, quindi, per larga parte dalle problematiche *ex* *ex* articolo 81 della Costituzione, sulle quali si è soffermato il ministro Tremonti: ovvero, la necessità di acquisire i dati finanziari sull'articolazione territoriale della spesa delle Regioni e degli enti locali, la simulazione matematica degli effetti dell'attuazione del federalismo fiscale e, in generale, le grandezze finanziarie mobilitate dal federalismo che stiamo progettando e l'impatto Lo hanno chiesto in modo perentorio il nostro relatore di minoranza, il senatore Vitali,

Ad una mia richiesta in tal senso, nella seduta del 13 novembre 2008, il presidente Baldassarri - che presiedeva appunto le tre Commissioni riunite - rispose testualmente: alla richiesta del senatore Legnini si associano anche gli altri membri delle tre Commissioni qui riunite. Quindi, tutti i componenti delle tre Commissioni, di maggioranza e di opposizione, fecero propria la richiesta di avere questi questi elementi quantitativi e numerici e di ottenere un quadro finanziario per valutare la portata dell'impianto legislativo in discussione.

un ampio consenso, non essendo sua intenzione costruire su indicazioni numeriche formule politiche che non corrispondono all'interesse del Paese».

dati e simulazioni in grado di valutarne *ex ante* la portata. L'esigenza di disporre dei dati quantitativi è ancora più forte ed evidente se si considera che il testo approvato dalle Commissioni riunite 1a,

ai principi di determinazione del costo e del fabbisogno standard, ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici di tutti i livelli di governo, al patto di convergenza, alla definizione dei servizi essenziali e non essenziali e quindi dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), alla disciplina tributaria locale, all'individuazione della Regione da utilizzare quale parametro per il finanziamento del fabbisogno corrispondente al livello dei LEP e ad altri punti. Eppure, non soltanto non ci sono stati forniti i dati nei termini evidenziati, ma la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario è rimasta invariata, come se tali importanti e sostanziali modificazioni fossero neutrali

ha smentito se stesso giacché poco più di un mese fa disse in Commissione che faceva propria la richiesta del nostro Gruppo di ottenere cifre, dati ed elementi di valutazione finanziaria. Quindi, signori Ministri,

Forniteci, dunque, i dati di cui disponete e, prima che l'Assemblea licenzi il provvedimento, saremo in grado di valutare la congruità, la coerenza e la completezza delle norme che dovremo approvare

in Commissione, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento. È una richiesta molto lontana da intenti dilatori o ostruzionistici - questo non c'entra nulla - ma dettata unicamente dall'esigenza di fare un lavoro completo ed il più possibile informato. Noi vogliamo questa riforma - lo abbiamo detto e lo ribadiamo - ma essa, così com'è, è senza rotta e non sarà capace di contenere tutte le istanze e le aspettative di cui avete inteso caricarla. Vogliamo essere sicuri che questo testo ci consentirà di coniugare più efficienza nell'erogazione dei servizi,

state bocciate - e, al contempo, ottenere l'accrescimento del grado di responsabilità dei vari livelli di Governo nei confronti dei cittadini. Avete il dovere di metterci nelle condizioni di farlo. Per questo vi chiediamo di accogliere la richiesta da noi avanzata, chiamando le Commissioni ad integrare il pur positivo lavoro svolto.

associate a quelle politiche del ministro Calderoli sugli aspetti di merito ed istituzionali che sono stati e sono oggetto di confronto parlamentare, confermano i dubbi, le perplessità ed i dissensi che noi abbiamo manifestato innanzitutto con la presentazione della pregiudiziale di costituzionalità, quindi con le questioni che abbiamo posto

di delega parlamentare, ma in sede di decreti delegati di attuazione, l'impegno che il Governo può assumere è solo ed esclusivamente di natura politica con le opposizioni, tenendo conto delle risultanze del dibattito parlamentare.

così come noi abbiamo prospettato nella pregiudiziale di costituzionalità, si tratta di un provvedimento che in questa fase può soltanto dare attuazione all'articolo 119, ma non può avere la presunzione di dare attuazione a quelle norme del Titolo V che hanno bisogno invece di una revisione costituzionale, com'è noto. Tanto è vero che il ministro Calderoli oggi ci parla dell'apertura ad un confronto sulla cosiddetta bozza Violante in tema di riforme costituzionali. Riteniamo altresì che non si possa costruire un assetto istituzionale e fiscale, ancorché privo di numeri e di coperture attuali, sulla scorta di funzioni amministrative tarate su una legislazione precedente all'entrata in vigore della riforma del Titolo V. Dal nostro punto di vista, infatti, la questione cruciale è anche questa:

consolidate rispetto alla legislazione anteriore alla riforma del Titolo V, che ha rivoluzionato il sistema delle competenze e quello dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali. La prova provata di tutto ciò è che, proprio per dare un minimo di copertura formale alla delega, si è inteso piazzare nel testo licenziato dalla Commissione l'individuazione esemplificativa di alcune funzioni fondamentali per i Comuni e per le Province, l'individuazione esemplificativa di alcuni livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l'indicazione, come clausola di stile e di chiusura, che tutte le funzioni sono quelle previste dalla legislazione vigente attualmente attribuite agli enti territoriali. la riforma del Titolo V non ha significato nulla, non ha prodotto alcuna rivoluzione sotto il profilo dell'assetto istituzionale dei rapporti.

dalla istituzione surrettizia con delega delle aree metropolitane senza che a ciò corrisponda lo scioglimento di un nodo fondamentale: che cosa si vuole fare delle Province. Si era detto che andavano soppresse; oggi non se ne parla più. Non si capisce in che termini e in che modo le aree metropolitane possano sovrapporsi (ovviamente per i territori interessati) alle Province esistenti. Tutto ciò innesta un ulteriore soggetto che ha autonomia di entrata e di spesa rispetto a quelli già previsti dalla legislazione ordinaria vigente. Queste ci sembrano, in verità, ragioni più che sufficienti per un ulteriore approfondimento. Pertanto, non possiamo che confermare, purtroppo, la nostra valutazione critica sul

un campionato o una riffa per cui vince chi è il più bravo secondo ciò che la cabina di regia decide. Quel fondo la Costituzione lo prevede per recuperare situazioni di disuguaglianza strutturale

neutralizzando l'attività amministrativa, delle disuguaglianze. In sostanza, quei territori e quei cittadini devono essere messi nelle condizioni di concorrere perché così prevede la Costituzione, che, precisamente al quinto comma dell'articolo 119, apposta risorse che lo Stato deve gestire

Presidente, ci inducono non solo a confermare le nostre perplessità, ma a sostenere, ancorché con motivazioni diverse, la richiesta che i colleghi del Partito Democratico hanno avanzato di non passare all'esame degli articoli perché riteniamo che questo sia il modo migliore per affrontare in maniera diversa e più efficace un tema che sta a cuore anche a noi, come a tutti i colleghi presenti in Parlamento.

Signora Presidente, la Lega Nord ovviamente voterà contro la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli e ritiene che sia assolutamente opportuno, nonché necessario, procedere sulla via della discussione di questo importante provvedimento. Un'importante riforma, che in Commissione abbiamo ampiamente discusso e condiviso. Con l'opposizione sono stati trovati numerosi punti di convergenza ed è proprio questo che vorremmo far rilevare all'Assemblea. Ad esempio, lo stesso presidente Morando, la cui competenza

possibile presentare tabelle compiute che vadano a quantificare l'effetto finale di questa riforma. Ma questo è nella logica delle cose.

Ciò che è importante, quindi, è l'aspetto procedurale. Come è stato detto, la risposta è sostanzialmente procedurale e nei meccanismi di controllo messi in campo, anche in questo caso prendendo i suggerimenti, condivisi nel merito, dell'opposizione, con la creazione di tutti questi organismi *ad* *hoc,* che avrannoil compito non solo formale, ma sostanziale di intervenire nella valutazione dei decreti delegati. La risposta quindi è soprattutto procedurale, ma la risposta, cari colleghi, è anche e soprattutto politica. Basterebbe una considerazione banale: abbiamo il terzo debito pubblico del mondo con l'attuale sistema di uso delle risorse. La Lega ritiene che sia il caso di cambiare e penso che ci sia poco da dire sul fatto che attualmente l'efficienza nell'uso delle risorse non è la migliore possibile. Signora Presidente, onorevoli colleghi, a me pare inevitabile che un provvedimento come questo sollevi interrogativi che non possono trovare immediatamente una risposta definitiva e del tutto rassicurante. L'articolata e scrupolosa risposta fornita poc'anzi dal ministro Tremonti ha messo in luce l'estrema complessità della materia che stiamo trattando anche implicitamente riconosciuto l'esigenza di cifrare puntualmente le singole norme, ma di cifrarle nella sede propria, che è quella dei decreti delegati. In altre circostanze è stato detto che per materie come questa prima vengono i numeri e poi le scelte. Stamane il ministro Tremonti ci ha detto invece, in maniera credo politicamente più intensa, che prima vengono le scelte e poi vengono i conti, fermo restando il fatto che, se i conti non dovessero tornare, si ritornerà sulle scelte. Quanto alla complessità della materia, io vorrei ricordare qui, per comune consapevolezza, l'esperienza relativamente modesta ma significativa delle Regioni a statuto speciale del nostro Paese. Dal 1948 la Sicilia e la Sardegna dispongono per statuto della compartecipazione all'IVA e all'IRPEF. Ebbene, solo per concordare le quote spettanti alle Regioni e allo Stato, i tavoli Stato-Regione hanno impiegato nel caso della Sardegna 60 anni, nel caso della Sicilia molto di meno, 59. Ora, davanti a tali difficoltà, che nel caso del federalismo fiscale si moltiplicheranno per molte volte, il ricorso alla legge delega appare per certi aspetti un danno, per altri invece un vantaggio. È un danno perché noi facciamo di fatto una riforma di estrema importanza con uno strumento legislativo che riduce di molto l'intervento del Parlamento nel processo legislativo. È un vantaggio perché con i decreti delegati e con i dispositivi che sono stati messi in essere per rafforzare i pareri del Parlamento la materia può essere affrontata e risolta in maniera efficace. Lo ha detto il ministro Tremonti, lo ripeto anch'io. Siamo di fronte ad una legge ordinaria, ma di estrema importanza, perché incide sulla Costituzione reale. E a noi è ben chiaro che nelle sue più minute articolazioni la legge e i decreti delegati che le daranno sostanza dovranno scrupolosamente osservare e rispettare l'articolo 5 della Costituzione: l'unità e la indivisibilità della Repubblica, che equivale all'unità e alla indivisibilità della Nazione. Il federalismo fiscale è un mezzo, ma l'unità della Nazione è un fine e questo fine è per tutti irrinunziabile. La Regione - diceva don Sturzo - nella Nazione, non contro la Nazione e neppure a prescindere dalla Nazione. In qualche modo - concludo, onorevoli colleghi - il voto favorevole che noi daremo al provvedimento conterrà una qualche riserva, che è nella attesa dei decreti delegati che dovranno dare forma definitiva al federalismo fiscale. Quindi, si tratta

sul parere rafforzato che questo provvedimento contiene. Allora, se così stanno le cose, e a me pare che così stiano, onorevoli colleghi,

e di mettere al più presto il Governo al lavoro perché poi il confronto si sviluppi in maniera più decisiva e in forme non più rinviabili sul terreno dell'elaborazione dei decreti e dell'emissione dei relativi pareri.

Il ministro Tremonti ci ha intrattenuto sul provvedimento in esame con una cortese verità accademica e ci ha illustrato le virtù dei sistemi olistici cui la complessità, l'interazione, la reciprocità finirebbero per determinare i caratteri di un universo indeterminato. Osservo solo di sfuggita che le grandezze economiche non sono un universo infinito e che il principio di indeterminazione classico funziona solo per la fisica delle particelle. Un ambito come quello, sia pure complicato e molteplice, del mondo economico è racchiudibile all'interno di un universo chiuso. del senatore Pisanu, osservo che i dubbi sul problema della costituzionalità non riguardano soltanto la questione dell'unità nazionale, ma soprattutto il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,

Il ministro Tremonti ha fatto una rassegna numerica: dodici tipi principali di tributi, cinque soggetti

Si potrebbero aggiungere alla rassegna numerica tre tipi di ambiguità che si rintracciano nell'intervento del Ministro: un'ambiguità di rilievo costituzionale, perché nel suo intervento affida la consistenza costituzionale del provvedimento ad una pura questione di fiducia nella volontà politica del Governo e della maggioranza; una forma di ambiguità politica, perché fa appello al fine, al cammino comune e ai passi da compiere, senza spiegare il mezzo, lo strumento; un'ambiguità logica, perché l'appello alla procedura condivisa contrasta con la prassi che vediamo negli ultimi tempi, una prassi di impoverimento dei Comuni nel momento in cui gli si sottraggono risorse e gli si promette un aumento futuro delle potestà.

Dichiaro aperta la votazione.

il senatore Legnini ha ragione a ricordare che in Commissione i Presidenti ed i membri della maggioranza hanno detto più volte, compreso il sottoscritto, che questo provvedimento aveva bisogno di una base di dati corretta. Non ha detto, però, il senatore Legnini che, in quella stessa sede, il presidente Baldassarri ed altri membri, contrariamente alle reiterate richieste del senatore Lusi,

e sui fabbisogni standard, quei conteggi sarebbero stati del tutto fuori luogo. La maggioranza si è impegnata, sin dall'esame in Commissione, a chiedere al Governo entro il primo anno, al momento dell'emanazione del primo decreto, di svolgere un lavoro serio per mettere a disposizione di tutti una base di dati corretta e significativa. quello che il ministro dell'economia Tremonti ha ripetuto qui questa mattina, facendo giustamente proprio l'impegno emerso in Commissione. Questo, per

Presidente, poiché il senatore Baldassarri ha fatto delle affermazioni abbastanza gravi, vorrei invitarlo, per rispetto della verità dei fatti, a controllare il verbale della seduta della Commissione a cui mi sono riferito (credo si tratti della seduta del 13 novembre 2008), laddove, a precisa richiesta del sottoscritto che, ripeto, era stata in precedenza formulata da altri colleghi, egli disse essere d'accordo e di fare propria quella richiesta. Non ho mistificato alcunché. Se oggi, in modo postumo, il senatore Baldassarri intende giustificare un suo comportamento, un suo mutamento di orientamento politico è libero di farlo, ma non può dire a me

perché non mi fido mai fino in fondo (e lo dico per corretta informazione dei senatori che non erano in Commissione e anche per sua corretta informazione),

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni riunite per il disegno di legge in titolo, premesso che l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica, che la disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza e nel corso dell'esame in Commissione è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie, che costituiscano un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei principi di federalismo fiscale; rilevata, pertanto, l'opportunità di procedere tempestivamente nelle conseguenti misure di revisione costituzionale e di innovazione legislativa; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Quanto all'articolo 2, commi 3 e 4, il parere è favorevole a condizione che siano introdotte alcune modifiche. In merito alla consultazione delle autonomie, affinché siano precisati gli effetti dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sia regolando il caso di una mancata intesa sia attribuendo al Governo un onere di motivazione per il possibile esito difforme del procedimento di legislazione per un'interpretazione che possa dare all'intesa la qualità di un presupposto assolutamente necessario e vincolante. Circa i pareri parlamentari, dovrebbe essere assicurata la simmetria tra quello della Commissione bicamerale e quelli delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario sotto l'aspetto degli effetti di un mancato parere nei termini di legge, ovvero della possibilità per il Governo di adottare comunque i decreti legislativi. Per le ragioni appena esposte si esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.715 e 2.750, mentre il parere è di nulla osta su tutti gli altri emendamenti con le osservazioni seguenti che rilevano altrettante anomalie: il 2.521, il 2.523 il 2.87 prevedono pareri parlamentari sottoposti al voto delle Assemblee e pareri parlamentari vincolanti su schemi di decreto legislativo; il 2.81 prevede più pareri parlamentari da parte di più organi bicamerali; il 2.520 postula una modificazione dei Regolamenti parlamentari, già prevista ma non ancora realizzata e, inoltre, ribadisce il carattere assolutamente necessario dell'intesa in sede di Conferenza unificata; il 3.1, al comma 3, prevede l'integrazione di un organo parlamentare, sia pure a effetti limitati ma con componenti estranei alle Camere; il 3.502 affida ai Consigli delle autonomie locali un ruolo non previsto dalla Costituzione (articolo 123)». previsto dalla Costituzione (articolo 123)». « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

di lavorare congiuntamente e in modo trasparente sugli stessi. I dati sono necessari e possibili decreto per decreto. Non è neanche richiesto dalla Costituzione sul testo della delega. Preciso in modo più chiaro perché forse non sono stato chiaro prima: la legge delega di attuazione del sistema di riforma di riforma regionale della Repubblica italiana, quindi un impianto generale assoluto, fu fatto senza valutazioni di impatto, presupponendo che quelle erano necessarie e fattibili a valle nei singoli provvedimenti attuativi. Lo stesso è avvenuto per la legge Bassanini e per tutte le grandi deleghe di questa Repubblica. I calcoli si fanno nel luogo giusto e, noi speriamo insieme a voi, nel modo giusto, cioè decreto per decreto. Nell'insieme complessivo la garanzia della tenuta è data dalla Costituzione, dalla norma che prevede l'equilibrio sociale e territoriale e dall'altra norma, pur importata dall'esterno, che impone l'equilibrio di bilancio in conformità con gli impegni europei.

anni non caratterizzati da particolari criticità economiche o sociali per l'Italia. Detto questo, se la domanda è più ampia - non: «Cosa vuol dire meno due punti?», ma: «Dove siamo e cosa succede?» - la premessa era stata: siamo in terra incognita. Siamo dentro una crisi che non ha precedenti nella storia recente. La combinazione tra la globalizzazione e la meccanica anche dell'informazione sono due novità assolute rispetto alle crisi precedenti. Ci siamo presentati in campagna elettorale con la formula «una crisi che arriva e che si aggrava», e questo è avvenuto nel marzo del 2008. Sappiamo bene che c'è la crisi.

Nell'attuazione del federalismo terremo fortemente conto di questo vincolo esterno e della differenza che c'è tra fare una riforma in un contesto normale e farla in un contesto di crisi. Sarà obiettivo del Governo evitare che l'attuazione della riforma costituisca un fattore di intensificazione o di prolungamento della crisi, ma anche questo oggetto sarà della discussione che faremo insieme, decreto per decreto.

l'intenzione di sopprimere il comma 2 per un motivo abbastanza preciso. Il disegno di legge in discussione vuole introdurre una riforma organica del finanziamento di Regioni ed enti locali che è fondamentalmente ispirato a principi di solidarietà, perequazione delle risorse, superamento della spesa storica, affermazione dell'autonomia e del riconoscimento del valore della responsabilità. questi principi non possono essere ristretti alle sole Regioni a statuto ordinario. Il comma 2, invece, prevede una sorta di deroga per le Regioni e le Province autonome.

**Il Senato non approva.**

riferiti all'articolo 2, la Presidenza chiede ai senatori Zanda e Poli Bortone di non insistere sui rispettivi emendamenti 2.521, 2.523 e 2.87, poiché tali emendamenti intervengono su materia coperta da riserva di Regolamento parlamentare o non sono conformi al modello di delegazione legislativa prevista dall'articolo 76 della Costituzione. La Presidenza, conformemente ai precedenti, non potrebbe infatti che dichiararne l'inammissibilità. Comprendo peraltro il senso delle proposte in questione, per cui la Presidenza ne consentirà comunque l'illustrazione, pur con questa richiesta.

«attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione». L'emendamento 2.500 propone che tali parole siano sostituite

parlamentare bicamerale che dovrà seguire l'attuazione del provvedimento nella fase dell'emanazione dei decreti delegati. Tremonti, se ce ne fosse stato bisogno, ha lui stesso oggi rafforzato le ragioni per cui questo emendamento era stato proposto. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un provvedimento di delega molto ampia e naturalmente è indefinito il numero dei decreti delegati,

palesemente sproporzionato rispetto all'ampiezza della delega e all'indeterminatezza dei principi che l'hanno definita. Mi spiace che il Regolamento del Senato non consenta di mantenere

anche sugli assetti istituzionali del federalismo fiscale, vorrei sintetizzare la nostra opinione come è contenuta in una serie di emendamenti a questo articolo. Lo faccio ora per ragioni di brevità, anche al fine di evitare di intervenire sui singoli emendamenti. Il punto centrale da cui partiamo è che non si può fare una riforma fiscale

e che costituiscono la vera rivoluzione della riscrittura dell'articolo 117. Infatti, l'articolo 117 dice che la funzione legislativa viene esercitata

e le altre in cui vige il principio della legislazione concorrente, che è diverso da quello disciplinato dalla vecchia formulazione dell'articolo 117, perché i principi fondamentali che si riserva lo Stato su tali materie hanno

normativa e legislativa alle Regioni anche in queste materie. Se così è, e tale è l'assetto costituzionale previsto dall'articolo 117, è chiaro che tutte le funzioni collegate alle materie che sono oggetto di legislazione concorrente (posto che la potestà regolamentare su questa materia è di competenza esclusiva delle Regioni) e tutte le materie che riguardano

nessuno pensa ad una scorciatoia. Il superamento della spesa storica sotto il profilo del trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali o comunque il superamento del concetto della spesa storica come metodo per l'amministrazione della cosa pubblica è assolutamente condiviso. Non condividiamo, invece, il modo in cui viene definito nel testo il concetto di costo e di fabbisogno standard. Infatti, l'unico elemento a cui è agganciato e che è certo nella delega (il resto è aria fritta)

che significa depurarlo dai costi dell'inefficienza della pubblica amministrazione, e un altro conto è non calcolare nel costo standard quei costi che sono il frutto del deficit infrastrutturale delle diverse situazioni di mercato. Un'impresa che svolge una prestazione nei confronti di una pubblica amministrazione del Sud sconta certamente due limiti: il primo è quello del costo del trasporto e il secondo è quello dell'accesso al credito.

anche il criterio di ripartizione del fondo perequativo; tuttavia il concetto di aliquota standard non viene definito nella delega. Allora, tutto ciò fa sì che il sistema centrale attraverso cui si definisce il riparto delle risorse, ivi compreso il sistema riguardante il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, si fondi su tale elemento. Pertanto, abbiamo proposto di temperare il criterio del superamento della spesa storica,

però, che non si può non comprendere nel concetto di costo standard anche l'oggettiva differenza territoriale che impone alle imprese, al sistema del credito e così via costi diversi, che comunque devono essere sopportati sopportati dalla pubblica amministrazione che, non avendo coperto il differenziale da risorse pubbliche, dovrà ricorrere all'autonomia impositiva; dovendo ricorrere al prelievo fiscale locale, ovviamente con il sistema delle addizionali determinerà

locali. Quando si ridistribuiscono le risorse (e su questo sono d'accordo), si ridistribuiscono di fatto anche i poteri. La Commissione, così come prevista nel testo licenziato dalle Commissioni riunite, è transitoria resta in vigore fino alla durata del periodo di adozione dei decreti attuativi. Quindi, tutta la fase di controllo parlamentare permanente esce da questo binario.

consentire al Parlamento di dare un indirizzo permanente nell'allineamento tra le funzioni e le risorse correlate.

al Parlamento e allo Stato. Queste funzioni pertanto non possono essere delegate, perché sono costituzionalmente riservate al Parlamento e allo Stato,

per un'urgenza evidente, quella di sveltire i tempi e rendere più certi i tempi della riforma. Questo emendamento sarà ripetuto in altri casi.

del ministro Calderoli e soprattutto del ministro Tremonti. Stiamo definendo un impianto di nuove modalità di finanziamento, che deve essere presidiato da principi e indirizzi tali da consentire che si dia effettivamente e concretamente attuazione ai principi costituzionali di tutela e salvaguardia delle funzioni che vengono riconosciute e trasferite ai livelli territoriali, regionale e locale. Questo è definito Ciò che è meno definito e meno rassicurante è la strumentazione e tutto l'impianto di accompagnamento che devono assecondare il processo per realizzare l'obiettivo. Mi riferisco, in particolare, al tema della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, con particolare riferimento ad una tipologia

è facilmente o abbastanza agevolmente ormai quantificabile. Questo tema è molto più complicato con riferimento all'assistenza, materia sulla quale non ci sono parametri fortemente raffrontabili, livelli e tipologie di servizi da sviluppare. Da questo punto di vista, allora, il passaggio dalla spesa storica al costo standard senza aver completato il quadro di riferimento di che cosa si deve individuare come tipologia di prestazioni, come vanno apprezzate e quantificate non dà assolutamente garanzia.

del patto di convergenza: affermati i principi e trovato il motore di riferimento e di regolazione, le cose potrebbero funzionare. Quello che manca, però, è una disamina puntuale che va inserita nei principi all'articolo 2, come noi proponiamo, di come si arriva a definire

la sede del patto di convergenza dovrebbe cercare di cercare di rendere armonico con le esigenze di compatibilità della finanza pubblica, graduando il processo evolutivo del sistema affinché tutti si allineino progressivamente ai livelli standard individuati. Se mancano questi due presupposti, mancano due parametri fondamentali dai quali non può che discendere tutto l'impianto successivo. Altrimenti il rischio è che si proceda

previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

poco coordinati tra loro sul piano degli adempimenti e della formalità, come pure delle tutele delle garanzie previste dallo statuto dei diritti del contribuente. Quest'ultimo

Il ministro Tremonti ha affermato che la titolarità, l'autonomia e le modalità del prelievo attengono ai principi della democrazia ed io credo che il tema della territorialità abbia proprio questo tipo di attinenza. infatti costituisce l'elemento in base al quale la titolarità delle imposte erariali è dello Stato e, conseguentemente, quelle imposte costituiscono un elemento essenziale per il finanziamento delle competenze e dei servizi propri dello Stato, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali dei cittadini e tutte le Ebbene, questo finanziamento, che avviene con imposte dedicate, ma anche, per quello che riguarda i territori più deboli, con la perequazione, deve avere un chiaro governo da parte dello Stato, in quanto garante dei diritti diritti fondamentali dei cittadini e delle pari opportunità e innalzamento delle condizioni di vita dei diversi territori.

in quanto stabilisce che la territorialità è unicamente collegata ai tributi regionali e locali e alle compartecipazioni. Perché questa sottolineatura è così importante? Perché abbiamo ben presente che cosa conteneva il modello legislativo previsto dalla Regione Lombardia, Lombardia, nonché come viene presentato alla pubblica opinione il tema del federalismo: ognuno tenga quello che produce sul proprio territorio; così viene letto nella *vulgata* corrente, con laconiugazione di un federalismo assolutamente egoista,

così come si è verificato via via, iniziando dal primo testo del Governo, ma soprattutto nel testo oggi in discussione in Aula, nel quale effettivamente ritengo sia stato chiarito ed acquisito qual è il senso della territorialità.

che attiene alle diverse caratteristiche dei nostri territori e in particolare alle zone più disagiate, tra cui cito la montagna e le isole minori. Ritengo quindi essenziale che venga accolto questo emendamento, che mi rendo conto può apparire come una duplicazione, ma mette il punto definitivo

abbiamo detto più volte che non siamo d'accordo sul fatto che costo e fabbisogno standard si rapportino e parametrino esclusivamente

inseriamo un altro elemento di indeterminatezza e di caratteristica generica, che è il «normale esercizio». Ho difficoltà a farmi spiegare dai colleghi che cosa sia il «normale esercizio delle funzioni pubbliche». 2, lettera *e)*, stabilisce che le risorse che vanno a copertura integrale delle funzioni

effetti critici per quanto riguarda l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore della sanità, dove già sono stati definiti, e provo difficoltà a constatare che siano stati applicati con criteri omogenei nelle venti Regioni d'Italia.

di poter intervenire in dichiarazione di voto

e l'emendamento 2.53, perché assorbiti rispettivamente da altri emendamenti che saranno posti

bisogna anche assumere il gettito generato dalle risorse naturali da valorizzare in un quadro di solidarietà e di federalismo, per compensare le limitazioni d'uso e i mancati usi alternativi del territorio. Tale misura peraltro è stata oggetto in altre circostanze di

Il solo riferimento alle basi imponibili ed aliquote appariva peraltro riduttivo. Dall'altra parte, volendo tenere aperta la possibilità di intervenire salvo compensazioni, è apparso opportuno non limitarla allo Stato, come pure di circoscriverla ai soli tributi attribuiti. Questa è la nostra proposta emendativa.

Signor Presidente, l'emendamento 2.55 intende risolvere un problema annoso che si trascina dal lontano 2000,

parte delle accise derivanti dal fatto che determinati comuni erano sede di impianti per lo stoccaggio e la produzione del petrolio, benzine e derivati. È noto che, laddove insistono queste strutture industriali, provocano una serie di problemi alla comunità che riguardano la qualità della vita, il trasporto, la salubrità dell'aria, l'eccesso di polveri sottili, quindi una serie di considerazioni che devono essere tenute presenti quando parliamo di federalismo, perché si possa effettivamente mettere a fuoco e valorizzare l'impianto di questa legge per tutta Italia, poiché allo stato risulta che soltanto per la Sicilia essa ha avuto effetti positivi ed è stata applicata. In tutte le altre Regioni, laddove insistono raffinerie e quant'altro, la suddetta legge non ha trovato applicazione. Quindi chiediamo che, con l'introduzione della normativa che riguarda il federalismo, venga applicato l'articolo 113 della legge che ho citato,

2.715 e 2.750, che corrispondono alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere favorevole sul testo proposto dalle Commissioni riunite. L'emendamento 2.715 precisa gli effetti dell'intesa in sede di Conferenza unificata, regolando il caso di una mancata intesa e attribuendo al Governo l'onere di una motivazione per il possibile esito difforme del procedimento di legislazione delegata rispetto ai contenuti della stessa. Vi sarebbe infatti un dubbio di compatibilità costituzionale per un'interpretazione che possa dare all'intesa la qualità di un presupposto assolutamente necessario e vincolante.

Presidente, avevo chiesto al presidente Chiti

settimana presenterà al Consiglio dei ministri la Carta delle autonomie locali. Un'iniziativa sicuramente positiva, parere è grave che, a distanza di una settimana, si presenti al Consiglio dei Ministri un testo che avrebbe dovuto essere propedeutico alla discussione in corso in questa Aula e che avrebbe chiarito

soprattutto i Comuni e gli enti locali in genere a più bassa capacità fiscale.

ricordando che questo testo viene presentato già nel frontespizio come applicativo dell'articolo 119 della Costituzione.

però tutta l'impostazione del provvedimento è improntata alla distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali.

Si dice con chiarezza: con la perequazione delle capacità fiscali. Ora, io ho provato a dialogare, perché devo dare atto che

*aa)* previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali,

questa perequazione debba avvenire attraverso il fondo perequativo o attraverso una perequazione delle capacità fiscali. Lo Stato cioè darebbe la possibilità ai Comuni più poveri

quali saranno le funzioni fondamentali e in quale campi occorrerà garantire i livelli essenziali delle prestazioni significa chiedere un voto senza sapere con chiarezza e precisione per che cosa si vota.

Tranne che non si voglia dire che la cultura, ministro Calderoli mi consenta, sia soltanto la sagra del maiale. Vi sono alcuni enti locali che vivono alimentando attività culturali anche in ordine ai beni culturali che possiedono e ciò rappresenta uno strumento di crescita e di sviluppo per le comunità locali. locali. In quell'elenco provvisorio poi non compaiono neppure l'infanzia e i minori, il che significa che la lotta alla devianza minorale, fondamentale nei Comuni, viene completamente relegata nelle funzioni non fondamentali che non abbiamo ancora capito bene come devono essere finanziate e con quali strumenti concreti ed operativi.

tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo finanziano integralmente le normali funzioni del Comune, cioè la stessa dicitura della Costituzione, senza specificare se riguardi quelle riferite alla lettera della Costituzione; le funzioni pubbliche sono dell'uno e dell'altro tipo. Nell'emendamento si chiede l'applicazione del costo standard a funzioni di cui non

però se lei avrà un po' di tempo disponibile - cosa che credo assai difficile - e andrà a vedere come quel principio viene poi declinato operativamente, si renderà conto che tutta l'impostazione del disegno di legge è nella distinzione tra le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali.

un parere contrario da parte del relatore e del Governo senza neanche, per esempio, prospettare, come avrei preso in considerazione, la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno di indirizzo, di criteri, perché la questione insiste sul tema su cui ci siamo intrattenuti.

avere qualche rassicurazione che il meccanismo procede secondo una sequenzialità logica e che la forfetizzazione o le macrocifre e i macroaggregati non sostituiscono l'individuazione di finanziamenti legati ad una valutazione di

specifica competenza, perché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle tipologie è una competenza assegnata alla legislazione nazionale.

debba operare nel pieno rispetto all'articolo 53 della Costituzione, che - com'è noto - invoca il principio della progressività delle imposte. Questo è il senso dell'emendamento,

per l'ovvia ragione che viene fatta salva l'autonomia degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale negli articoli successivi, con possibilità per quelle Regioni, nella loro autonomia, di valutare tale questione.

le prerogative - come è noto al senatore Cuffaro - sono tali che le nostre possibilità di intervento sono limitate.

siciliana e non una legge ordinaria. Diversamente, approveremmo leggi che non si tengono in piedi.

Qui si sta introducendo un elemento nuovo che vale per le Regioni a statuto ordinario. Per la tutela del nostro Statuto non dobbiamo perdere un'occasione. Mi pare obiettivamente che quel che desideravano i

nelle garanzie statutarie un elemento di vantaggio e non di limite a questa previsione

quando precisano queste eccezioni che riguardano le Regioni a Statuto speciale, di completare sempre il testo o l'intervento, perché è una didascalia costituzionalmente garantita, «e le due Province autonome di Trento e Bolzano». La cosa sembra implicita, ma se non si precisa si creano inutili allarmismi, temendo che le due Province autonome, che hanno prerogative identiche o superiori,

Presidente, richiamo di nuovo l'attenzione sia del Presidente della Commissione, che del ministro Calderoli: stiamo approvando una norma che riguarda il federalismo e mai come in questo caso deve ritornare agli enti locali - quindi ai Comuni, alle Regioni e così via - la potestà di verificare la possibilità di trattenere le accise sul territorio, laddove ci sono impianti industriali di raffinazione che provocano enormi disagi alla popolazione. Ricordo al Ministro e alla Lega che nella battaglia che facemmo nel 2000 per la legge n. 388, che cito in questo emendamento,

ha trovato applicazione soltanto in una realtà della Sicilia e non vedo perché non si possa procedere oggi, in materia di federalismo fiscale, ad applicarla su tutto il territorio nazionale.

Senatrice Sbarbati, lei ha pienamente ragione nell'intervenire e nel chiedere chiarimenti, ma è nel diritto del Governo intervenire o no. Ciascuno in quest'Aula assume delle posizioni e si assume le proprie responsabilità in merito ai contenuti, alle proposte,

**Il Senato non approva.**

poiché esso interviene su una materia delicata qual è quella delle risorse umane utilizzate nelle autonomie locali, quindi i dipendenti. Questo tipo di provvedimento crea di per sé una strana situazione

Non vorremmo che all'interno del costo standard, all'improvviso, una strana autonomia concessa ad ogni ente locale provocasse una rivendicazione in negativo sul personale, per cui si guardasse al futuro rispetto alle funzioni e si ritornasse agli anni '80 rispetto al contratto di lavoro dei dipendenti delle autonomie locali. Noi abbiamo ottenuto in quegli anni il contratto collettivo nazionale; ridare una singola autonomia che non faccia riferimento magari al secondo livello di contrattazione, alla professionalità, alla produttività o all'organizzazione del lavoro, che è altro rispetto all'autonomia concessa *tout court* e rispetto al contratto,

non dà attuazione all'articolo 118 con il trasferimento di funzioni e, tanto meno, vengono trasferite materie che richiederebbero un intervento costituzionale.

ma diventi dipendente regionale, posso dire che non cambia alcunché in quanto la funzione resta allo stesso livello. Se qualcuno vuol mettere all'ordine del giorno che l'intervento (da parte mia condiviso, ma io con il lavoro non c'entro alcunché), per esempio la contrattazione di secondo livello, possa avvenire anche a livelli inferiori a quello statale, ma in senso positivo non negativo, perché non posso negare quello che non

cosa diversa da una regolamentazione sul trasferimento di personale e sul regime dovuto al trattamento del personale; stiamo parlando di contrattazione collettiva. Nel momento in cui si dà autonomia ad ogni singolo ente locale di fare contrattazione collettiva significa ritornare a fare in modo che ogni Comune definisca i suoi contratti in base all'autonomia impositiva. Questo recita il dettato. Rispetto a tale situazione, credo che vada fatta una considerazione, perché il rischio reale - così come avviene in Europa

di fissare tali principi. Quindi non si sta dando alcun potere o ruolo al di sotto che non sia quello che lo Stato decida in relazione a questo.

che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determini aumento della pressione fiscale statale, regionale e locale.

perché non è solo il senatore dell'opposizione che lamenta tariffe predatorie ma un rappresentante del Governo, l'onorevole Roberto Castelli. Rispetto a questo non si può far finta di nulla. Non si può regalare ai capitani coraggiosi

*(PD)*. Signor Presidente, parlo al sesto giorno di sciopero della fame mentre l'onorevoli Beltrandi, oltre a non mangiare da sette giorni, occupa la Commissione di vigilanza da giovedì scorso.

RAI. Chiedo di sapere quando verranno rese note le motivazioni di questa gravissima decisione perché bisognerà che qualcuno, che ancora un minimo pratica la legalità delle nostre istituzioni, vi si opponga o se non altro prenda in considerazione la possibilità di

ci si è assunta la responsabilità di tenere al di fuori della legalità costituzionale una Commissione che deve non soltanto rinnovare il Consiglio di amministrazione della RAI, ma anche adottare tutta una serie di misure relativamente alle campagne elettorali prossime venture e all'accesso all'accesso ai nostri programmi radiotelevisivi di tutta una serie di organizzazioni. I radicali italiani hanno presentato una denuncia alla quale la RAI ha risposto che ha risposto che in mancanza della Commissione di vigilanza tutto ciò non può essere deciso. La Commissione non esiste. Non soltanto si è in spregio agli obblighi della nostra Costituzione, ma si sta facendo anche un torto a tutti coloro i quali, attraverso il servizio pubblico, possono fare informazione relativamente alle proprie iniziative. La domanda comunque resta e vorremmo sapere quando verranno pubblicate le motivazioni relativamente alla gravissima decisione presa stamani. **Per

il problema non c'è, perché non è un atto ripetibile, in quanto i verbali sono a testimonianza di quanto accaduto. Gradirei che certi fatti non si verificassero più in futuro; per quanto mi riguarda è tutto abbastanza chiaro. Sul secondo motivo per cui ho chiesto la parola, Presidente,

Io non cito più il numero e la data delle interrogazioni; chiedo la cortesia agli Uffici di verificare le interrogazioni presentate dal sottoscritto con altri colleghi senatori che non hanno ricevuto mai risposta, sia che siano state sollecitate sia che siano state doverosamente e scolasticamente

nelle pagine genovesi ha usato lo sgarbo di pubblicare i nomi di tutti i senatori eletti in Liguria (cosa che mi onora, essendo fra questi), perché una solerte giornalista, venerdì

Questo giornale ha pubblicato ieri un articolo in tutta evidenza, secondo il quale ben 16 senatori eletti in quella Regione, fra cui il sottoscritto, non avrebbero risposto alla domanda di un cittadino (simulato, visto che era una giornalista che cercava di capire quanto fossimo bravi o non bravi

come il sottoscritto, lo abbia indicato. Simili episodi non fanno piacere a nessuno di noi senatori, indipendentemente dalla

affinché tutte le autorità e gli organi dello Stato intervengano in difesa innanzi tutto della magistratura, che ha condannato

è però particolarmente grave nella giornata di oggi perché su «la Repubblica» leggo un articolo di Claudio Tito con dichiarazioni virgolettate di Ministri, a cominciare dal ministro Calderoli, che prendono posizione

alle due questioni non legate alle interrogazioni che sono state sollevate dal senatore Perduca, come ha già detto il senatore Ceccanti, è stato espresso

Battisti non si chiuda e possa essere estradato in Italia. Condividiamo il giudizio dato dal Presidente della Repubblica per primo: il nostro è uno Stato di diritto ed in uno Stato di diritto, nella reciprocità dei rapporti tra i vari Stati, chi è condannato all'ergastolo per omicidio